finestra"). La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha definito all'unanimità il calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'8 febbraio prossimo. Per quanto concerne le votazioni previste per oggi pomeriggio, in particolare i voti qualificati sulla riforma dell'articolo 5 del Regolamento, la Presidenza, in relazione a disagi nel traffico aereo, valuterà - se del caso - l'eventualità del rinvio delle votazioni ad un momento in cui l'Assemblea sia in condizioni di *plenum*. Oltre agli argomenti previsti dall'ordine del giorno di oggi pomeriggio, restano confermati per questa settimana gli altri punti già stabiliti: il decreto‑legge recante abrogazione di una norma in materia di illeciti contabili, fin da domani mattina, fin da domani mattina, con eventuale seguito nel pomeriggio, nonché le dimissioni presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga, al primo punto della seduta pomeridiana di domani. Si aggiunge inoltre, sempre in settimana, l'avvio della discussione generale del disegno di legge sul disagio abitativo, che proseguirà nella seduta antimeridiana di martedì 6 febbraio. La discussione sulle mozioni e altri strumenti di sindacato ispettivo sull'ampliamento della base USA di Vicenza, già prevista per giovedì 1o febbraio, avrà inizio alle ore 9, anziché alle ore 9,30, e si concluderà con il voto entro la fine della seduta. A tal fine i tempi sono stati ripartiti per complessive cinque ore, comprensive di illustrazioni, repliche e dichiarazioni di voto finali. Nella settimana successiva, dal 6 all'8 febbraio, saranno discussi il disegno di legge sul disagio abitativo, le dimissioni reiterate da senatori facenti parte del Governo (queste ultime nella seduta pomeridiana di mercoledì 7 febbraio), nonché, nella mattinata di giovedì 8, la mozione Andreotti ed altri per l'istituzione di una Commissione speciale sui diritti umani e ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto sull'opportunità di ricostituire anche in questa legislatura il Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Ricordo che per l'approvazione delle modifiche al Regolamento, l'articolo 64, primo comma, della Costituzione e l'articolo 167, comma 5, del Regolamento prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato, cioè 162 voti. Al testo unificato dei documenti II, nn. 5 e 6, é stato presentato l'emendamento 1.1, a firma del senatore Stiffoni e altri, sottoposto all'esame della Giunta nella seduta del 19 dicembre 2006.

i due documenti contengono proposte, sostanzialmente identiche fra loro, di modifica dell'articolo 5 del Regolamento del Senato, che interviene a disciplinare l'elezione di coloro

Mi rivolgo a tutti i colleghi e con particolare calore ai colleghi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale.

Non indugio nell'illustrare le relative modalità di votazione - anch'esse ben note - limitandomi a sottolineare come uno degli effetti che le stesse normalmente determinano consista nell'assicurare rappresentatività a tutti i Gruppi politici costituenti l'Assemblea, attraverso l'assunzione - da parte di almeno un esponente degli stessi - dell'uno o dell'altro incarico di quelli facenti capo alla Presidenza. Ho detto «uno degli effetti che le stesse normalmente determinano» perché in realtà un'inversa situazione si è - e si potrebbe dire eccezionalmente - determinata in occasione della formazione della Presidenza della legislatura che è in corso. Ciò è quanto è argomentato dal Gruppo di Democrazia Cristiana-Partito Repubblicano Italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia, il quale, ricordando come la propria costituzione abbia avuto luogo sostanzialmente sin dall'inizio della legislatura, sebbene qualche giorno dopo che l'Assemblea ebbe ad eleggere i componenti della Presidenza, obietta come, proprio e in qualche modo solo per tale specifica ragione, nessuno dei propri aderenti abbia potuto essere chiamato ad alcuno dei sopra citati incarichi. Ma, in realtà, non di questo - in sé - si duole il detto Gruppo, quanto del fatto che da ciò derivi, come conseguenza, la sua esclusione dalle attività e dalle attribuzioni che il Regolamento riserva, attraverso l'articolo 12, al Consiglio di Presidenza: la sua non partecipazione, in altre parole, all'attività di amministrazione del Senato. Credo di poter dire che il rilievo ha carattere oggettivo nella sua fondatezza. Come del resto non diversamente è nel diverso caso che è illustrato nella proposta avanzata con il documento II, n. 5, d'iniziativa del senatore Formisano. Questi, Presidente del Gruppo Misto, ricorda la circostanza (anche in questo caso in qualche modo eccezionale, rispetto a quella ordinarietà che prima sottolineavo) determinatasi nel momento in cui si costituì il Gruppo per le Autonomie, con conseguente - direi naturale - adesione allo stesso da parte della senatrice Thaler Ausserhofer. Ciò avvenne quasi alla fine del mese di maggio dello scorso anno, dopo che alla stessa già era tuttavia assegnato l'incarico di senatore Questore e, quindi, di componente del Consiglio di Presidenza, con conseguente perdita di rappresentatività nell'ambito dello stesso da parte del Gruppo Misto, cui la senatrice aveva all'inizio aderito, non risultando ancora costituito il suo Gruppo. Fattispecie, dunque, distinta rispetto a quella prima illustrata, in relazione all'ulteriore documento in esame, ma assolutamente identica quanto alla situazione che si è determinata e che è in atto. Come sostanzialmente identiche sono le soluzioni che risultano proposte e che la Giunta per il Regolamento ha esaminato nella sua penultima seduta, con conseguente assegnazione dell'incarico - cui ora adempio - di riferire all'Assemblea. Il percorso proposto è, in definitiva, il seguente. Il Gruppo rimasto privo di rappresentatività nel Consiglio di Presidenza, e che senta la necessità di rimuovere tale condizione, deve sottoporre la questione al Consiglio di Presidenza stesso, il quale provvede "con delibera a seguito di richiesta". La richiesta da proporre è quella dell'elezione di ulteriori senatori Segretari e la delibera che il Consiglio può assumere è quella della relativa indizione, perché la stessa abbia luogo, limitatamente ad ulteriori due senatori Segretari, e non più di due. Il Presidente del Senato dà attuazione alla detta delibera del Consiglio di Presidenza secondo le modalità indicate dal comma 2-*ter*, congegnato in maniera tale da inevitabilmente determinare l'elezione a Segretario di un senatore che abbia aderito al Gruppo richiedente in ragione di quanto prima detto. Detto ciò, non può sottacersi come un eventuale problema potrebbe certamente nascere ove i Gruppi richiedenti siano più di uno (e superiori a due) e se tutte le relative richieste risultino accolte dal Consiglio di Presidenza. Il meccanismo di voto è infatti tale da determinare che, in tale caso, una o più delle richieste possano rimanere non soddisfatte per effetto della limitazione di cui prima dicevo. Ma non è questo un problema che trova oggi attualità. Resta ferma, secondo il mio avviso, l'opportunità di verificare la necessità di prospettiva di una complessiva riconsiderazione dell'intero sistema di governo del Senato, in una direzione che sia influenzata da molteplici presupposti logici e di razionalità e che sia anche rispondente alla necessità di fornire adeguate e legittime risposte di matrice più spiccatamente politica (tra cui vi sono, senz'altro, quelle che possono essere ora trovate, all'insegna dell'attualità), ma credo di dover conclusivamente dire che la soluzione proposta, e che ho descritto, è oggi senz'altro tale da determinare il risultato auspicato e la stessa dovrà pertanto essere adottata ove sia condiviso il perseguimento di tale risultato. risultato. Come lei ha annunciato, signor Presidente, risulta proposto un emendamento da parte del senatore Stiffoni e di altri senatori, sul quale mi indicherà quando dovrò intervenire. La Giunta per il Regolamento ha introdotto una disposizione, che i colleghi trovano nel documento a loro disposizione (che è novità rispetto ai due documenti originariamente presentati), che individua l'entrata in vigore della nuova disposizione del Regolamento, ove la stessa fosse adottata, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si tratta di un'aggiunta di cui è assolutamente evidente la virtuosa finalità, che è quella di fissare, in maniera esatta e non discutibile, il momento dell'entrata in vigore della nuova

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi per discutere su un'iniziativa volta a modificare il Regolamento interno al Senato, o meglio ad adeguare lo stesso ad una specifica esigenza di rappresentatività che è emersa durante questa legislatura. Dobbiamo infatti ricordare che il Consiglio di Presidenza, previsto e regolamentato nella sua composizione e nelle sue funzioni dal Regolamento stesso, è il massimo organo di riferimento del Senato, non solo sotto il profilo relativo allo svolgimento dell'attività legislativa o all'attività prettamente politica, quanto e più allo svolgimento delle quotidiane e straordinarie attività amministrative del Senato stesso. In base al Regolamento, infatti, il Consiglio di Presidenza delibera il progetto di bilancio del Senato; delibera le sanzioni nei confronti dei senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato; approva i Regolamenti interni all'amministrazione; adotta tutti i provvedimenti relativi al personale, sia sotto il profilo gestionale sia concorsuale. funzioni, si può affermare che esso sia l'organo che provvede alla gestione dell'intero Senato sotto il profilo amministrativo‑regolamentare e, tramite il suo Presidente, è il garante del buon andamento

la volontà e gli interessi di ogni singolo senatore. Non poter partecipare al Consiglio di Presidenza significa, infatti, non prendere parte alla vita amministrativa del Senato stesso e a quelle decisioni che consentono di mandare avanti l'organizzazione nel suo insieme. Allo stato attuale dei fatti, non viene rispettato lo spirito che infonde il Consiglio ed il Regolamento, volto a ricercare e a garantire un insieme di equilibrio tra le sue varie componenti necessarie.

Io affermo che tale reale intenzione, sottesa nella norma regolamentare, non è attualmente rispettata poiché all'inizio di questa legislatura sono rimasti, per vicende differenti, esclusi due Gruppi, costituitisi secondo le norme del Regolamento stesso e i quali non hanno potuto vedere eletti, all'interno del Consiglio di Presidenza, un proprio rappresentante, impedendogli in tal modo di manifestare la volontà dei propri componenti e determinando quindi una distorsione e una diversità nel funzionamento del Consiglio stesso.

non ha potuto veder eletto un suo componente. In base a tale considerazione, ho chiesto, tramite questa mia proposta, una modifica al Regolamento del Senato e chiedo all'Assemblea l'approvazione della stessa per ripristinare un giusto equilibrio.

Signor Presidente, farò solo poche considerazioni per motivare il mio personale dissenso sulla proposta di modificare l'articolo 5 del Regolamento del Senato. L'istituto del Consiglio di Presidenza trova fondamento nell'articolo 63 della Costituzione e l'articolo 64 ne disciplina il funzionamento. Il Consiglio di Presidenza ha funzioni importanti nel campo della direzione amministrativa, ma compiti ben limitati in merito allo svolgimento dei lavori parlamentari e alla libertà di dibattito in Assemblea. Non voglio in questa sede affrontare il problema delle funzioni né tanto meno i riflessi rispetto al sistema elettorale.

Operare con rammendi, come direbbe il senatore Manzella, non è un buon metodo. Qui non è in discussione il principio di difesa delle minoranze, un principio riconosciuto dalla nostra tradizione parlamentare, ma qualcosa d'altro. Intanto, viene modificata una norma che dal 1988 ad oggi ha subito ben quattro modifiche (nel 1988, nel 1993, nel 1999 e nel 2001), una norma «elastico» che muta a seconda delle circostanze. Partiamo dal primo punto. Il Gruppo Misto aveva fatto le proprie scelte, era autorevolmente rappresentato nel Consiglio di Presidenza. Non vi può essere una rappresentanza variabile nel Consiglio di Presidenza a seconda delle convenienze. Questa modifica regolamentare aprirebbe il fianco ad altre modifiche. Il principio per cui le minoranze devono essere rappresentate si consolida attraverso un'antica tradizione parlamentare, intesa ad assicurare la massima obiettività ed imparzialità nel funzionamento di questo organo collegiale dell'Assemblea, di rango costituzionale. Ma qui non è in discussione la difesa delle minoranze, ma la proliferazione la proliferazione delle poltrone. In tal modo si determinano le condizioni per ulteriori frammentazioni della rappresentanza parlamentare. Che cosa avverrebbe - mi domando - se nei Gruppi maggiori si determinassero rotture con conseguenti proliferazioni dei Gruppi parlamentari? Si aumenterebbe ulteriormente il numero dei Segretari di Presidenza. Sappiamo bene, Presidente, come sono andate le cose! Il Gruppo per le Autonomie è stato funzionale agli interessi della maggioranza, non rifletteva un risultato elettorale, è diventato un *escamotage* per superare le difficoltà della maggioranza nelle Commissioni parlamentari. Tutto ciò si è riflesso nella rappresentanza del Gruppo Misto che oggi si vuole assecondare con un rimedio peggiore del male. Questa modifica al Regolamento, dunque, non convince.

Il Gruppo Misto, che richiede una rappresentanza, è già rappresentato nell'organo più squisitamente politico, che è la Conferenza dei Capigruppo. Capigruppo. Inoltre, ha già contribuito con le sue scelte agli assetti istituzionali, così come sono stati definiti immediatamente dopo l'elezione con la costituzione del Consiglio di Presidenza. Ritengo che già trova rappresentanza in sede di Conferenza dei Capigruppo, certamente una sede di rappresentanza di interessi più squisitamente politici. Esprimo, quindi, il mio personale dissenso ad una proliferazione che nuoce al buon andamento dei lavori e alle ragioni di rappresentatività. Qui non siamo in presenza della nascita di nuovi movimenti politici. Le elezioni sono la fotografia politica di riferimento alla quale ci si deve ancorare. Per queste ragioni, esprimo forti perplessità sulla scelta che si sta operando, che non convince per ragioni istituzionali prima ancora che politiche. Ritengo che non si possano introdurre modifiche regolamentari ad uso di accordi politici.

stiamo esaminando una modifica all'articolo 5 del Regolamento che è orientata a riespandere il principio di rappresentanza in seno al Consiglio di Presidenza, modificando quanto il Senato aveva già deciso all'inizio della passata legislatura. La modifica consiste, sostanzialmente, nell'aumentare il numero dei Segretari da otto La norma regolamentare originaria, che adesso dobbiamo reintrodurre, era infatti ispirata chiaramente alla interpretazione più estensiva del principio di rappresentanza, inteso quale diritto

che ha fissato in modo rigido a otto il numero dei senatori Segretari, ammettendone l'elezione con voto limitato a quattro, aveva in maniera evidente anteposto al principio di rappresentanza dei Gruppi quello di rappresentanza delle coalizioni di maggioranza e di opposizione. Ricorderete che all'epoca era stato argomentato che in tal modo il Consiglio di Presidenza avrebbe meglio rispecchiato nella sua composizione la maggioranza politica espressa dall'Assemblea. Quella scelta, in realtà, non si è dimostrata adeguata per due ordini di ragioni. La prima ragione risiede nel mancato adeguamento complessivo dei Regolamenti parlamentari ai risultati derivanti dal mutamento introdotto nel sistema politico dal sistema elettorale maggioritario. Infatti, senza un adeguamento complessivo - che peraltro, voglio ricordare, nella passata

La seconda ragione ha invece carattere storico, perché il Senato ben hapresente come la nuova legge elettorale del 2006 abbia mutato l'impianto maggioritario del nostro meccanismo elettorale in senso più proporzionalista, favorendo quindi la proliferazione dei Gruppi parlamentari. In questo senso e a maggior ragione, appare oggi naturale ripristinare il vecchio principio di rappresentanza nella sua accezione più ampia, giacché non farlo significherebbe in qualche modo comprimere le prerogative di partecipazione di una porzione significativa delle forze politiche rappresentate in Senato. Delresto, l'analisi delle funzioni oggi attribuite al Consiglio di Presidenza è un elemento

elenca le attribuzioni del Consiglio di Presidenza, evidenziandone le funzioni di gestione dell'istituzione, a cominciare - lo voglio ricordare a titolo soltanto di esempio - dalla predisposizione del progetto di bilancio del Senato, l'approvazione del Regolamento della Biblioteca, la nomina del Segretario generale, l'approvazione di Regolamenti interni e così via. Le considerazioni svolte inducono a qualificare il Consiglio di Presidenza quale sede deliberativa e cruciale strumento di garanzia, giustificando, per la sua composizione, modalità che valorizzino al massimo il principio partecipativo. In definitiva, le istanze di modifica all'articolo 5 che stiamo esaminando e che la Giunta per il Regolamento ha approvato debbono ritenersi il frutto, in qualche modo obbligato, del nuovo assetto del sistema politico italiano quale si è determinato in conseguenza della riforma elettorale approvata nella scorsa legislatura e delle caratteristiche quasi di «bipolarismo proporzionale» che ha assunto il nostro Parlamento. In questo senso, voteremo a favore della modifica approvata dalla Giunta per il Regolamento. *(Applausi

con l'emendamento 1.1 si intende riscrivere completamente l'articolo 5 del Regolamento del Senato. La sostanza della modifica proposta sta nello statuire che ogni Gruppo esistente alla data di costituzione delle Commissioni permanenti ha diritto, per la propria rappresentanza nel Consiglio di Presidenza, ad avere un proprio Segretario e ciò per un contatto più diretto dei Gruppi con la struttura che gestisce il Senato. Qualcuno senz'altro potrà obiettare, e l'ha già fatto, che già tra i Vice presidenti vi sono componenti dei Gruppi e che pertanto vi è un'adeguata rappresentatività. Vorrei però evidenziare che i Vice presidenti hanno un ruolo istituzionale che i Segretari non hanno e che, appunto per questa ragione, è evidente che vi è stato, al momento della loro elezione, un raccordo tra Camera e Senato per l'inserimento di parlamentari rappresentativi delle varie realtà di maggioranza e di opposizione. Signor Presidente, i Vice presidenti svolgono una funzione, i Segretari un'altra. Faccio altresì presente che alla Camera, ed è un discorso di omogeneità ci dovrebbe essere tra la Camera e il Senato, i Segretari sono ben 16, in rappresentanza di tutte le componenti politiche, al di là dei Gruppi costituiti; componenti politiche che hanno una consistenza numerica molto limitata, ben al di sotto del numero minimo previsto dal Regolamento della Camera, che ne prevede 20. Vorrei ricordare che come Segretari di Segretari di Presidenza alla Camera vi sono rappresentanti di Gruppi che hanno la consistenza di 16, 6, 19, 18, 14, e anche 10 Signor Presidente, innanzitutto l'emendamento 1.1 non è assolutamente in contrapposizione ai testi proposti dai colleghi

proporrei, mi rivolgo a tutti ma specificatamente ai colleghi Capigruppo, di procedere in questo modo: per prima cosa chiediamo il parere del relatore sull'emendamento presentato dal senatore Stiffoni ed altri,

le votazioni su entrambi i testi, sia l'emendamento che il testo illustrato dal senatore Caruso, Caruso, si svolgano nella seduta di domani. Questo per la ragione molto semplice che entrambe le votazioni devono avvenire con procedimento elettronico ed è richiesta la maggioranza di 162

È un argomento che non ritengo convincente. Il senatore Stiffoni mira a dire che il Segretario piuttosto che il Vice presidente hanno ruoli e *status* diversi all'interno del Consiglio di Presidenza. Ciò non corrisponde al vero, nel senso che è assolutamente ovvio che il Vice presidente svolga funzioni che gli sono proprie come è altrettanto ovvio che il Segretario svolga funzioni che gli sono proprie, ma nel momento in cui entrambi partecipano a quella che il nostro Regolamento definisce la Presidenza, vale a dire l'organo di gestione dell'Assemblea. Tutt'affatto diversa è la loro posizione, assolutamente paritaria - si distingue solamente quella del Presidente del Senato - nel diverso ambito, viceversa, del Consiglio di Presidenza, cui sono attribuiti compiti tutt'affatto diversi. Quindi, rinnovo la richiesta al senatore Stiffoni di ritirare l'emendamento 1.1; diversamente esprimo parere contrario. La richiesta di ritirare l'emendamento non è solo segnata da ragioni di cortesia nei confronti del collega - che comunque è dovuta - ma anche dal fatto che il collega con la propria proposta pone una questione, che anch'io mi sono permesso di illustrare, di sfondo, rispetto alla necessità, all'opportunità forse, che si provveda a riconsiderare la funzione e la composizione del Consiglio di Presidenza, individuandolo non già come un soggetto derivato dalla Presidenza e integrato da un rappresentante per ciascun Gruppo solo limitatamente ad alcune sue funzioni, ma, viceversa, come soggetto cui è affidata l'amministrazione del Senato e quindi con delle specificità

Mi permetto di ripetere che esso non è assolutamente in contrasto con il testo presentato dagli altri due colleghi; anzi, dà la possibilità a tutti i Gruppi presenti in Senato di avere una propria rappresentanza, al di là di figure che sono state elette, magari alla carica di Vice presidente, che hanno - ripeto - un ruolo istituzionale di altro tipo rispetto a quello che hanno i Segretari propriamente detti. Ribadisco il concetto prima espresso; non voglio fare raffronti tra un ramo del Parlamento e l'altro, mi sembra tuttavia che alla Camera questo tipo di rappresentatività di tutti i Gruppi sia stato esteso anche a Gruppi che hanno una consistenza numerica assolutamente non conforme a quanto sarebbe previsto per la costituzione di un Gruppo. In effetti, sei deputati certamente non fanno parte di un Gruppo alla Camera; ciò nonostante è stato concesso di avere un loro rappresentante all'interno del Consiglio di Presidenza.

intervengo per esprimere la mia perplessità su quanto sembra essere deliberato

anche a quelli nei quali un membro riveste già un'alta carica del Senato, di poter essere presenti in Consiglio di Presidenza con un Segretario d'Aula.

che d'altra parte rispecchiano l'ampia riflessione fatta in sede di Giunta per il Regolamento. Poiché si tratta di far fronte a due circostanze abbastanza eccezionali ed il provvedimento contiene un ampliamento limitato del numero dei componenti

la cortesia di sapere se queste votazioni avverranno domani, prima o dopo l'argomento già posto all'ordine del giorno perchè, se avvengono prima, il rischio di mancanza della maggioranza assoluta è molto alto.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 novembre 2006, l'Assemblea ha deliberato di rinviare la discussione ad altra seduta.

*(Ulivo)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho letto accuratamente le due relazioni presentate dal collega senatore Berselli perché riguardano due procedimenti penali diversi. Le relazioni sono sostanzialmente speculari nel senso che ripropongono le stesse motivazioni per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti e la proposta della Giunta al termine dell'attività svolta. La prima questione riguarda la ricostruzione del fatto storico, che è pacifico, ed è stato esemplarmente illustrato nelle due relazioni del senatore Berselli. è soltanto un'indicazione riportata nelle due relazioni e ripetuta anche poco fa in Aula relativa al fatto che la Giunta per le elezioni avrebbe all'unanimità dato indicazione per il non accoglimento delle richieste della magistratura per la prosecuzione del procedimento penale. Si tratta di un'unanimità da un punto di vista formale, perché era l'unanimità dei presenti. Nel momento in cui la Giunta ha votato, vi era una maggioranza che voleva decidere nel senso del ricorso presentato dal senatore Iannuzzi;

non avendo i numeri, ha deciso di uscire dall'Aula in cui si teneva la riunione della Giunta. Sono rimasti dunque i senatori dell'attuale opposizione politica, che hanno votato all'unanimità. La mia illustrazione si presenta come un intervento in qualità di rappresentante del Gruppo Ulivo all'interno della Giunta e si limiterà all'indicazione, il più possibile asettica, dell'accusa formulata dall'autorità giudiziaria di Milano ed a quelle che sono le impostazioni di stretto diritto per quanto riguarda tali situazioni. Per quanto riguarda la prima richiesta di deliberazione, avanzata dal Tribunale di Milano il 16 gennaio 2006, essa riguarda i parenti - moglie e figlio - del sindacalista assassinato Domenico Geraci che, in un articolo pubblicato, era stato accusato di aver fatto da tramite tra la mafia e ambienti di sinistra. L'articolo letteralmente prosegue dicendo: «Si disse perfino che Geraci, un *boss* camorrista, era su quello stesso aereo in cui viaggiarono da Palermo a Roma Luciano Violante e Giovanni Brusca». L'articolo risale al 10 ottobre 2002 e questa è l'accusa di diffamazione formulata sulla base della querela presentata dalla moglie e dal figlio del sindacalista, indicato appunto come molto discusso e che avrebbe fatto da tramite tra la mafia e ambienti di sinistra. La seconda questione riguarda, invece, una querela che è stata presentata

all'unanimità di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

che fa ritenere che situazioni di questo tipo non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, viene detto nella relazione dello stesso senatore Berselli che tale tesi della Corte costituzionale non è condivisibile. Viene detto altresì che si comprendono le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale ad adottare tale indirizzo però ribadito che tale orientamento non può essere ritenuto esaustivo dell'area in cui opera la guarentigia dell'insindacabilità.

non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro di una delle due Camere: nesso funzionale che, nel caso di dichiarazioni rese *extra moenia*, presuppone che queste ultime possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari. «Indipendentemente dall'eventuale contenuto diffamatorio delle dichiarazioni stesse, il compito di questa Corte è quindi limitato alla verifica se esse, ancorché rese fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare: se costituiscano, cioè, espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno».

all'imputato la commissione di illeciti specifici e puntualmente localizzati al di fuori del territorio di competenza. Per quanto riguarda, in particolare, dichiarazioni rese attraverso la stampa,

che riporta, poi, gli stessi concetti che ho citato poco fa riferendo della relazione del senatore Berselli. In questa ultima sentenza del novembre 2006, la Corte costituzionale ripete: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'articolo 21 della Costituzione». Conclude la Corte sul punto dicendo: «In tale prospettiva, va anche disatteso l'assunto del Senato, secondo cui «l'attività di parlamentare e giornalista, dalla quale ha avuto origine l'articolo *de* *quo*, [può] essere considerata ormai come parte della più ampia attività (*rectius*, funzione) di politico ed espressione - per quanto atipica - del relativo ruolo istituzionale»: questa Corte ha, infatti, già ritenuto in sé irrilevante (al fine di affermare la sussistenza dei presupposti dell'insindacabilità) la qualifica rivestita dal membro del Parlamento rispetto all'esercizio di diritti o di doveri

La situazione che si presenta ora a quest'Aula è molto semplice: c'è una giurisprudenza (ricordata dal relatore Berselli) concorde da vari anni

per l'organo parlamentare nel suo insieme di proporre, qualora non sia d'accordo con la giurisprudenza della Corte costituzionale, delle norme diverse a migliore delucidazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Presidente, senatrici, senatori, va ricordato che la Giunta delle

Direi che è stata anche affrettata la decisione di decidere, non consentendo, appunto, in quella sede, un approfondimento e una discussione. Noi del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea arriviamo a questa discussione in modo sofferto. Come si sa, infatti, anche in epoca in cui le immunità nel nostro Paese sembravano a taluni la copertura dal malaffare, abbiamo difeso un principio garantista.

garantisce, appunto, la libertà d'espressione; in particolare, la garantisce alle opposizioni, soprattutto in relazione ad una funzione del ruolo del parlamentare di fronte a gangli complessi della nostra società. Penso a quanti hanno denunciato, anche grazie all'articolo 68, i gangli dei rapporti del potere mafioso, del suo controllo sulla società e, attraverso questo uso, hanno anche contribuito a far crescere una coscienza civile e

ammesso - va detto e riconosciuto - del tutto limpidamente nel confronto con la Giunta, ha un rapporto retributivo con «Il Giornale» e quindi un vero e proprio rapporto

seppur legittimamente, non essendo stata consentita appieno una discussione all'interno della Giunta. Abbiamo deciso, dicevo, soffertamente di aderire alla conclusione che

mezzo stampa. Siamo in presenza proprio di quella provocazione. Riteniamo, però, che sia più alta la necessità di difendere la possibilità di libertà e di scelta di opinione, anche di fronte a queste provocazioni. Per questo voteremo sull'indicazione che qui è stata data.

un passaggio anche importante per il Parlamento. Credo che attestarsi sulla lettura acritica e formalistica della giurisprudenza della Corte sia un atteggiamento del tutto erroneo, che ritengo dobbiamo responsabilmente modificare, soprattutto di fronte a situazioni - lo ricordo ai colleghi - che non hanno quei connotati di strumentalizzazione della prerogativa parlamentare finalizzata a vere e proprie attività diffamatorie. Ritengo invece la prerogativa possa essere invocata per difendere la libertà di espressione di un membro del Parlamento, colleghi, che di questi argomenti, di questi temi, di queste vicende si è sempre occupato, che siede in quest'Aula e la cui presenza è pertanto riconosciuta sotto questo profilo per le battaglie che ha combattuto sui temi più in genere della giustizia.

La prima potrebbe essere burocratica se non considerassimo che la Corte, quando enuncia questi princìpi - invito i colleghi a riflettere su questo passaggio - lo fa non nella sede di di verifica di sindacato della legittimità di una legge, ma nella sede di conflitto di attribuzione, laddove il fatto che emerge volta per volta è l'elemento che può determinare una decisione piuttosto che un'altra. Purtroppo in passato non fa onore all'Aula e al Parlamento - spesso, ripeto, si è usata la guarentigia dell'articolo 68 in maniera strumentale. Su questi episodi la Corte ha espresso le sue linee linee di condotta. Però, qui siamo in ipotesi completamente diverse e credo che il Parlamento e quest'Aula farebbero cosa estremamente positiva se rivendicassero una loro dignità istituzionale affermando che l'articolo 68 è una garanzia non per il singolo parlamentare, ma per l'intero Parlamento. In secondo luogo, la lettura, in linea con le sentenze della Corte in materie comunque diverse da questa, sarebbe ipocrita perché se il collega Iannuzzi, ben consapevole della giurisprudenza della Corte, avesse voluto dare seguito a quella giurisprudenza, avrebbe potuto presentare un minuto prima un'interrogazione parlamentare, redigere il suo articolo e vederlo pubblicato un minuto dopo, per essere sicuramente coperto dall'immunità dell'articolo 68. Allora, il collega Iannuzzi questo non solo non l'ha fatto, ma - se ne deve dare atto - non ha neanche voluto farlo, perché - ci ha dichiarato in Giunta - si sarebbe sentito diminuito nella sua dignità personale e professionale se avesse seguito questo percorso. Se vogliamo allora dare una risposta a queste vicende, credo

il Parlamento e quello che vi è al di fuori del Parlamento. Le garanzie dell'articolo 68 sono preziose; sono le ultime garanzie che rimangono ai parlamentari e credo che ogni volta che si delibera su queste, occorra fare un'approfondita riflessione e non fermarsi all'apparenza della situazione che in quel momento dobbiamo giudicare. PRESIDENTE.

Presidente, il collega Casson ha esposto, per conto del nostro Gruppo, i termini della questione. Lo ha fatto perché tutti i colleghi del nostro Gruppo, ma anche dell'Assemblea, potessero esprimere il loro voto D'altro canto il relatore, nel raccontare i fatti, ha espresso in maniera altrettanto puntuale le premesse di questa nostra decisione. C'è un periodo che riassume chiaramente la questione: «I querelanti, rispettivamente figlio e coniuge di Domenico Geraci, lamentavano che il loro congiunto, ucciso nell'ottobre 1998, fosse stato definito - in un inciso dell'articolo a firma del senatore Iannuzzi, in cui si elencavano i delitti di cui si era accollato o meno la responsabilità il collaborante di giustizia Antonino Giuffrè - «un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra (si disse perfino che Geraci era su quello stesso aereo in cui viaggiarono da Palermo a Roma Luciano Violante e Giovanni Brusca)». I familiari, nella querela, rivendicavano la posizione di costante contrasto alla presenza condizionante della mafia "in molteplici settori dell'attività economica, politica ed ed amministrativa di Caccamo e non solo", esercitata da Domenico Geraci, dirigente provinciale dell'associazione sindacale UIL». Questi i termini della questione, che sono stati molto ben ripresi dal collega che ha illustrato la posizione giuridico‑istituzionale, senatore Casson. Tutti hanno ora la possibilità di votare secondo coscienza e di esprimere, con il loro voto, un assenso o un dissenso sulle decisioni della Giunta.

Senatore Casson, stiamo votando sulla prima delle questioni che è stata sollevata; successivamente voteremo sulla seconda e infine sulla terza, che riguarda il conflitto di attribuzione

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nella seduta antimeridiana del 23 novembre 2006, l'Assemblea ha deliberato di rinviare la discussione ad altra seduta. Chiedo al relatore, senatore Berselli, se intende intervenire.

nel senso che è identica la persona indagata, sono diverse le parti offese; la situazione procedimentale, giuridica è del tutto identica, nel senso che c'è stato un voto unanime dei presenti in Giunta per gli stessi motivi che sono stati indicati in precedenza, in particolare dal senatore Boccia. Per quanto riguarda la diversità della situazione, il capo di imputazione è chiaro e specifico: riguarda un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale», in data 23 ottobre 2003, e riguarda l'offesa della reputazione di alcuni magistrati della procura della Repubblica di Palermo, in particolare il dottor Caselli, il dottor Lo Forte, il dottor Scarpinato e il dottor Natoli, in relazione a situazioni che concernevano la Commissione antimafia, l'inizio del processo Andreotti e il fatto di aver messo «le mani sulla procura di Palermo» e a di avere insediato - così viene detto letteralmente - «il suo compagno di cultura giacobina e di ventura progressista Giancarlo Caselli». Le indicazioni che sono state fornite per la prima di queste relazioni sono identiche: si ripropone un conflitto tra il Senato e la Corte costituzionale, per quanto riguarda la valutazione delle norme di rango costituzionale, sia la Costituzione sia la legge costituzionale che riguarda l'articolo 68, primo comma, Quindi, mi riporto a quanto dichiarato pochi minuti fa a questo proposito, rappresentando che in questa situazione, come in altre situazioni recenti, già è stato affrontato dalla Corte costituzionale un conflitto tra l'autorità giudiziaria e il Parlamento, in particolare il Senato, che è stato risolto dalla Corte costituzionale a favore dell'autorità giudiziaria. In questa situazione di palese ed evidente contraddizione tra le due posizioni, sarebbe probabilmente più opportuno un intervento normativo a specificazione del contenuto dell'articolo 68 della nostra Costituzione.

elezioni e delle immunità parlamentari*. **Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano** con ricorso del 7 luglio 2006, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 15 febbraio 2006, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 9135/05 RGNR - 6693/05 GIP, pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 4 dicembre 2006, n. 420, depositata in cancelleria il successivo 14 dicembre e notificata al Senato il 17 gennaio 2007. Nella seduta odierna la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto. Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Con una deliberazione che riprendeva un deliberato della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari quest'Aula, nella scorsa legislatura, accertava l'applicabilità dell'esimente di cui all'articolo 68 al collega Iannuzzi rispetto ad alcuni fatti che gli venivano contestati. Quindi, ne conseguiva l'insindacabilità che è stata in qualche modo contestata dal GIP di Milano, che ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Rispetto al conflitto di attribuzione la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità. Siamo quindi nella fase nella quale, dopo l'avvenuta dichiarazione di ammissibilità, le parti devono comparire dinanzi alla Corte per sostenere le proprie ragioni.

non posso che prendere atto di un deliberato di questa Assemblea, che legittimamente si è espressa. Quella espressione di volontà ha radicato un convincimento riferibile all'articolo 68 che poi ha dato origine al conflitto. le indagini preliminari di Milano ritenga che il deliberato dell'Assemblea del Senato possa dar luogo a un conflitto e chieda quindi il vaglio e il giudicato della Corte costituzionale, noi dobbiamo stabilire adesso se è legittimo che il Senato possa rappresentare le ragioni che hanno determinato quel volto dinanzi alla Corte costituzionale. Anche se ho votato contro in quella sede, non posso che continuare a sostenere che il deliberato è stato assunto in maniera legittima e che quindi il Senato debba poter coltivare il diritto di difesa dinanzi alla Corte costituzionale. So già che molto probabilmente, per una giurisprudenza ormai consolidata che dovrebbe indurre quest'Assemblea a rivisitare l'articolo 68, probabilmente la Corte accoglierà il conflitto, ma questo non mi induce a ritenere che il Senato debba rimanere privo contenzioso. Ecco perché ho detto in Giunta questa mattina e adesso in Aula ribadisco che, a mio avviso, è necessario che il Senato coltivi le sue ragioni, tutelando i suoi interessi ribaditi con quella delibera legittimamente assunta.

registrazione dei nomi, le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere